che operano nel territorio italiano, prevista dall'articolo 31 della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2021. In particolare, il senatore interrogante sottolinea che alcune associazioni di categoria hanno espresso contrarietà a tale previsione normativa, lamentando la possibilità di un incremento del contenzioso con i consumatori e incertezza sulla procedura liquidatoria da seguire. Conseguentemente, sono stati richiesti chiarimenti all'applicazione temporale della norma ed è stata suggerita la proroga dell'entrata in vigore della nuova disciplina al 30 giugno 2024, anziché quella prevista per il gennaio del 2023 e quindi in corso.

sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese. L'Ivass ha sottolineato come l'estensione dell'obbligo di adesione anche alle imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea elimini il potenziale effetto discriminatorio a danno delle imprese italiane, nonché il rischio di alterare le dinamiche di mercato. Inoltre ha ricordato che in occasione dell'audizione alla Commissione X della Camera, svoltasi nel giugno 2022, è emersa l'adeguatezza del termine del 1° gennaio 2023, recepito poi nel testo normativo definitivo. Pertanto, la richiesta di proroga in questione sinora non ha ricevuto seguito. La nuova disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 per tutti i la richiesta di proroga in questione sinora non ha ricevuto seguito. La nuova disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2023 per tutti i sinistri successivi a questa data. L'Ivass ha ricordato altresì di aver emanato diversi provvedimenti atti a migliorare il funzionamento del sistema CARD, aggiungendo al primo meccanismo forfettario di calcolo del rimborso un successivo criterio di calcolo con incentivi e penalizzazioni, vedendo con favore ogni miglioramento del sistema che contribuisca ad aumentare l'efficienza complessiva del sistema. Sul tema, sollevato dal senatore interrogante, posso confermare dunque da parte del Ministero un monitoraggio dello stato di attuazione della disciplina in parola e sugli impatti tariffari della stessa sui premi assicurativi, al fine di valutare, ove necessario, di intraprendere possibili ulteriori iniziative per assicurare l'efficienza operativa del sistema, da un lato, e la tutela del consumatore, dall'altro.

sicuramente necessaria, per tutelare sia i consumatori, sia le imprese da un'indebita disparità di trattamento che si poteva verificare tra imprese italiane ed estere che non fossero dentro il sistema CARD.

un *broker* assicurativo che attivamente partecipa ai vantaggi della non applicabilità del sistema CARD alle imprese estere; e ci proveranno sempre tutti coloro che cercheranno di trarre un guadagno e un vantaggio dalla non applicazione del sistema CARD alle imprese estere. Ecco perché noi continueremo a vigilare. Giustamente, lei ha citato l'Ivass, che era infatti parte anche dell'interrogazione, affinché la corretta applicazione della normativa sulla concorrenza e l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 del sistema CARD possano garantire, da una parte, l'equa e leale concorrenza tra le imprese e, dall'altra, i vantaggi che i consumatori, quindi anche i cittadini italiani, hanno dalla corretta applicazione del sistema CARD. La ringraziamo quindi per la risposta e noi continueremo a vigilare affinché questo sistema non conosca deroghe o scorciatoie.

di cattura e stoccaggio di anidride carbonica, denominato CCS Ravenna fase 1, si rappresenta quanto segue. Il progetto in parola è riferito all'esecuzione di un programma sperimentale di cattura, trasporto e stoccaggio geologico di anidride carbonica (CO2), proveniente dalla centrale di Casalborsetti, per un volume pari a 25.000 tonnellate all'anno, con una durata d'iniezione pari a un massimo di due anni nel complesso di stoccaggio individuato dal livello esaurito del campo Porto Corsini mare Ovest, operante in forza della concessione rilasciata da ENI con decreto ministeriale del 18 giugno 1998 e prorogata, con decreto ministeriale del 5 aprile 2012, fino al 1° gennaio 2027. Innanzitutto, si specifica che il progetto è candidato ad avere lo *status* di progetto di interesse comune europeo, ovvero di far parte di quei progetti che potranno accedere al bando per l'ottenimento dei finanziamenti del Connecting europe facility, il fondo UE volto al potenziamento delle infrastrutture energetiche di trasporto digitali che, per il periodo 2021-2027, assegna al settore energetico un *budget* di 5,8 miliardi di euro. In particolare, in coordinamento con Air Liquide France Industrie, in collaborazione con ENI e Snam, in un'ottica di condivisione progettuale sovraterritoriale, CCS Ravenna fase 1 ha l'obiettivo di sviluppare, nell'area del Mediterraneo, infrastrutture per *import* ed *export* di CO2, ponendo al centro la città di Ravenna e, nello specifico, i giacimenti gas *offshore* in via di esaurimento in concessione ad ENI, che sarebbero trasformati in siti per lo stoccaggio di CO2 degli impianti industriali italiani ed esteri. L'intervento, pertanto, mira a contribuire alla rimozione delle emissioni, consentendo il trasporto e lo stoccaggio geologico della CO2 catturata dai punti di emissione industriali a un sito di stoccaggio *offshore*, atteso che il processo necessita di ulteriori autorizzazioni all'iniezione che, una volta presentate, verranno valutate alla luce della normativa vigente. L'istanza di autorizzazione all'esecuzione del programma è stata presentata al Ministero da ENI il 31 maggio 2021 e l'ufficio competente, a seguito della verifica dei requisiti tecnici e amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza stessa, ha dato corso al relativo *iter* autorizzativo, che ricade nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 162 del 2011, il quale, in attuazione della direttiva, stabilisce un quadro di misure volte a garantire lo stoccaggio geologico della CO2 in formazioni geologiche idonee. Con successive modificazioni sopramenzionato decreto legislativo, intervenute con il decreto-legge n. 76 del 2020, è stato ulteriormente disciplinato che l'autorizzazione venga rilasciata dal MASE, su parere del Comitato ETS (Emission trading territorialmente interessata, mediante un procedimento unico di conferenze di servizi, ai sensi della legge n. 241 del 1990, nel cui ambito vengono acquisiti gli atti di assenso di tutte le amministrazioni e ditte interessate. Inoltre, essendo il volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore alle 100.000 tonnellate, il predetto *iter* ha seguito una procedura semplificata, che non richiede l'interlocuzione con la Commissione europea, né gli adempimenti inerenti alla concorrenza, né pertanto l'assoggettamento a preventiva valutazione d'impatto ambientale. Ciò premesso, si rappresenta che è stata completata presso questo Ministero la procedura di rilascio dell'autorizzazione in parola, in linea con le risultanze favorevoli dell'attività istruttoria, nonché corredata delle prescrizioni espresse nel corso del procedimento, anche in seguito all'avvenuta emanazione, il 21 dicembre 2022, dell'atto d'intesa da parte della Regione Emilia-Romagna. È necessario specificare che il progetto finalizzato all'acquisizione dei dati tecnici ed economici atti a testare l'efficacia e la sicurezza dell'intero sistema di cattura e stoccaggio per un eventuale sviluppo su scala industriale e ulteriori ampliamenti relativi ai punti di prelievo connessi ad eventuali successive fasi del progetto saranno debitamente valutati, qualora sottoposti a istanza di autorizzazione dal punto di vista sia tecnico sia procedimentale.

della sua migliorata competitività in sede di valutazione economico-ingegneristica rispetto al passato. Inoltre, lo stesso Comitato ETS, in premessa al parere rilasciato per il progetto sperimentale oggetto dell'interrogazione, ritiene che, anche per effetto dell'aumento del prezzo ripresa l'attenzione per la tecnologia CCS da parte delle imprese interessate, quale strumento ausiliare per l'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. D'altra parte, risultano essere presenti nel mondo 21 impianti CCS in attività, 3 in costruzione, 17 in fase avanzata di sviluppo e 24 in fase iniziale. L'Europa, in particolare, annovera in proposito alcuni impianti in attività, segnatamente in Norvegia, e ha in previsione nuovi progetti, alcuni in stato avanzato di programmazione, altri ancora allo studio. Va rilevato infine come la normativa vigente in materia, a seguito delle modifiche normative, riconosca la rilevanza strategica della tecnologia CCS nel quadro della politica energetica ambientale del nostro Paese, proiettata verso la decarbonizzazione,

del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. In ultimo, riguardo alla sicurezza e alla sostenibilità economica del progetto presentato da ENI, si evidenzia ancora una volta che nel corso del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di autorizzazione sono stati accertati, oltre che i dati concernenti gli aspetti localizzativi, geologici e sismici, anche quelli relativi agli aspetti di sicurezza, attesa la comprovata competenza dei membri componenti la segreteria tecnica del citato Comitato ETS in rappresentanza dei Ministri coinvolti dagli istituti di ricerca. Atteso quanto esposto, il progetto in questione potrà eventualmente accedere a forme di finanziamento pubblico soltanto in relazione ai suddetti fondi europei, ovvero nel caso in cui venga inserito nella lista dei progetti di interesse comune europeo.

si continua a perseguire una strada di non decarbonizzazione veramente allarmante. Sono risorse che vengono sottratte alle nuove generazioni, ai nuovi lavori e alla sicurezza dell'ambiente e che vengono investite, al di là della transizione energetica,

sperimentazione su un territorio che penso abbia già dato tanto in questi anni. Abbiamo bisogno di investire e Ravenna è una città che ha il *know how* perfetto per capire, per affrontare per migliorare il suo percorso di transizione energetica. Purtroppo, però, invece di accelerare gli investimenti sulle fonti rinnovabili, si trovano gli spazi per indirizzare la nostra attenzione a livello di Governo

al termovalorizzatore ubicato in località Picchianti nel Comune di Livorno, si rappresenta quanto segue. Innanzitutto, è opportuno premettere che la competenza in materia di autorizzazione del citato impianto di trattamento dei rifiuti è in carico alle amministrazioni regionali, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso specifico, la Regione Toscana rappresenta che l'impianto in questione, gestito dalla società Aamps SpA, è stato autorizzato dalla Provincia di Livorno con autorizzazione integrata ambientale (AIA) del 30 ottobre 2007, con scadenza al 30 ottobre 2015 e successivamente prorogata al 30 ottobre 2023. Si rappresenta che la Regione Toscana ha emesso atti di modifica e aggiornamento dell'AIA nel 2017-2018 e infine nel 2020. Nell'aprile del 2021 la società Aamps SpA ha presentato ulteriore istanza di modifica dell'AIA ai sensi dell'articolo del testo unico ambientale (TUA), a seguito del quale la Regione ha rilasciato un provvedimento di aggiornamento, reintroducendo fra le attività le operazioni di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati, al fine di permettere che la frazione secca fosse destinata all'alimentazione del termovalorizzatore. Tuttavia, il 14 marzo 2022 gli uffici preposti della Regione, in forza dell'articolo 29-*octies* del TUA, che prevede il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle decisioni relative alle conclusioni sulle *best available technique* (BAT), e alla luce delle pubblicazioni relative alla decisione UE della Commissione del novembre 2019, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (le cosiddette BAT), hanno dato avvio a una specifica nota al procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA per l'adeguamento delle BAT citate. Le cosiddette BAT *conclusion* consistono nella sintesi delle migliori tecniche disponibili, comprendenti la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio necessario, i livelli di consumo, ovvero i valori limite di emissione e le altre condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione. Arrivata suddetta nota, pertanto, si sospendeva contestualmente il procedimento, in attesa che la società Aamps presentasse tutta la documentazione tecnica necessaria per il riesame dell'autorizzazione. In merito, la società che gestisce il termovalorizzatore ha presentato la necessaria documentazione, richiesta e sollecitata dalla Regione, in data 30 novembre del 2022. La Regione Toscana rappresenta altresì che, ad oggi, a seguito della pubblicazione dell'avviso pubblico, è in corso il procedimento di riesame dell'AIA. La Regione, inoltre, evidenzia come il progetto di riesame dell'AIA, presentato dalla società Aamps, si coordina con la condizione alla prosecuzione della funzione di impianto integrato dell'ambito territoriale ottimale (ATO) Toscana, oggi rappresentato dal termovalorizzatore, oltre il termine dell'entrata in completo esercizio della nuova tecnologia ad ossicombustione, ipotizzata alla fine del 2026, attesa la necessità di presentare un progetto di trasformazione e/o dismissione del termovalorizzatore in base all'attuale testo dell'AIA. La Regione specifica ancora che nella documentazione presentata emerge l'ipotesi di superamento dell'impianto esistente, in quanto la società Reti ambiente SpA ha approvato, con delibera dell'assemblea dei soci, il *masterplan* 2030 degli *asset* industriali, che consente l'importante progetto di costruzione di una piattaforma ad ossicombustione presso la discarica di Peccioli, nel Comune di Pisa, destinata a coprire le esigenze di trattamento finale dei rifiuti in tutto l'ambito territoriale dell'ATO Toscana-Costa. Nell'evidenziare come sia la Regione l'amministrazione competente per le attività di ricognizione degli impianti di trattamento dei rifiuti, compresa la decisione di realizzare ulteriori nuove infrastrutture o di determinare la chiusura di quelle esistenti, nell'ambito delle interlocuzioni tra il Ministero e gli enti territoriali interessati alla vicenda, sarà presa in considerazione ogni eventuale istanza che provenga dal territorio toscano, anche al fine di coadiuvare le istituzioni locali nella ricerca della migliore soluzione.

provengo. Questo è un caso che rispecchia anche la mancanza di una programmazione lungimirante, perché la città di Livorno sta vivendo un

Purtroppo qui siamo di fronte ad un caso nel quale, ad esempio, lato costa, si va incontro allo spegnimento di un impianto che sta garantendo produzione elettrica, quindi un utile per la società municipalizzata,

La tecnologia di questa parte del territorio è infatti ferma, sostanzialmente, all'utilizzo della discarica quale strumento per chiudere il ciclo dei rifiuti. Io lo chiamo il semiciclo, perché in realtà la discarica non chiude un bel niente e non fa che lasciare ai posteri il problema di una gestione la chiusura di questo impianto è frutto purtroppo di una visione ideologica pregiudiziale verso lo strumento della termovalorizzazione. Sappiamo benissimo che la raccolta differenziata è condizione necessaria, ma non sufficiente a completare quello che si chiama il ciclo dei rifiuti. Stiamo e state investendo risorse veramente

nell'inettitudine di alcuni amministratori locali, soprattutto quelli del territorio dal quale provengo, per l'indeterminatezza, l'incertezza e probabilmente anche l'ignoranza di una visione d'insieme che sta

a tonnellata per costo di smaltimento, con la chiusura del termovalorizzatore di Livorno essa certamente

cooperazione internazionale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, fornisco un'unica risposta alle interrogazioni 3-00034 della senatrice Camusso e 3-00059 della senatrice Gelmini. Il Governo italiano segue con grande preoccupazione quanto accade in Iran. Le notizie di esecuzioni e di gravissime e violazioni dei diritti umani nei confronti di giovani in custodia delle autorità, in violazione degli *standard* internazionali sui diritti umani, suscitano profondo sgomento. Il ricorso alla pena di morte per soffocare le proteste ha segnato un punto di non ritorno. Il Governo, in sintonia con il diffuso sentimento di indignazione della nostra opinione pubblica e della società civile, ha reagito immediatamente sia a livello nazionale sia in ambito europeo e multilaterale. A livello internazionale, il ministro Tajani ha convocato, il 28 dicembre scorso, l'ambasciatore iraniano a Roma, che allora non aveva ancora presentato le credenziali: un'iniziativa straordinaria adottata in raccordo con il Quirinale, resa necessaria dalla gravità della situazione. In quell'occasione il ministro Tajani, a nome del Governo, ha chiesto alle autorità iraniane, per il tramite dell'ambasciatore Saburi, di non procedere ad altre esecuzioni capitali; di fermare la repressione delle proteste e ogni violazione dei diritti umani dei manifestanti e di coloro che sono stati arrestati in connessione con le proteste; di adottare un atteggiamento improntato al dialogo con i manifestanti e all'ascolto della società, soprattutto di giovani e donne; di adottare un atteggiamento responsabile anche sul piano regionale. Il presidente Mattarella, nel ricevere le credenziali dell'ambasciatore iraniano l'11 gennaio, ha espresso la ferma condanna della Repubblica Italiana e la sua personale indignazione per la brutale repressione, le condanne a morte e le esecuzioni di molti dimostranti. Il nostro Paese - è giusto ricordarlo - è in prima linea per la moratoria universale sulle esecuzioni capitali in vista della loro abolizione ovunque nel mondo. Nel dicembre 2022 siamo passati da 123 a 125 voti a favore della risoluzione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite biennale sulla moratoria: un risultato importante, frutto anche di un lavoro di squadra con la società civile, in particolare con la Comunità di Sant'Egidio, Nessuno tocchi Caino e Amnesty International, con cui intendiamo continuare a collaborare e i cui rappresentanti ho incontrato personalmente. Come segnale di vicinanza alla popolazione iraniana, abbiamo incontrato alla Farnesina un nutrito gruppo di studenti iraniani in Italia. Sono stati accolti dalla collega Tripodi, su delega del ministro Tajani. Abbiamo ascoltato i racconti e le richieste dei giovani, esprimendo la profonda solidarietà delle istituzioni e dell'opinione pubblica italiane. Abbiamo ribadito la ferma condanna per le brutali azioni repressive condotte dalle autorità sui manifestanti, anche in ambito europeo, cosa che consente senza dubbio una maggiore efficacia d'azione. La nostra risposta è stata immediata e ferma. Abbiamo fatto ricorso allo strumento sanzionatorio inquadrato nel regime per violazioni gravi dei diritti umani già in vigore dal 2011. In occasione di consecutivi Consigli dei ministri degli affari esteri dell'Unione (del 17 ottobre, del 14 novembre, del 12 dicembre e del 23 gennaio), sono stati adottati quattro pacchetti di sanzioni contro enti e individui iraniani, responsabili della morte di Mahsa Amini e della repressione violenta delle proteste che ne sono seguite; stiamo lavorando ora a una quinta tornata. A queste misure si aggiungono le sanzioni approvate a ottobre e a dicembre contro individui ed entità iraniane per violazione dell'integrità territoriale ucraina, in relazione alla fornitura di droni iraniani alla Russia, utilizzati nel conflitto in Ucraina. Abbiamo incoraggiato un approccio improntato all'equilibrio e alla gradualità, per rendere lo strumento sanzionatorio credibile ed efficace. Nelle conclusioni adottate dal Consiglio affari esteri il 12 dicembre scorso è stata condannata senza mezzi termini la repressione violenta delle proteste da parte delle autorità iraniane. Il documento si sofferma su altre questioni di particolare sensibilità, dalla fornitura di droni a Mosca alle attività destabilizzanti nella regione. Sul programma nucleare, le conclusioni del Consiglio lasciano aperta la possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran. Ciò rappresenterebbe un risultato importante per il contrasto alla proliferazione nucleare e quindi per la stabilità regionale. Anche in ambito Nazioni Unite l'Italia ha sostenuto numerose iniziative. Abbiamo co-sponsorizzato la risoluzione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU adottata il 24 novembre, che ha istituito una missione internazionale indipendente per indagare sulle violazioni dei diritti umani in relazione alle proteste. La situazione dei diritti umani in Iran sarà nuovamente all'attenzione del Consiglio diritti umani alla fine del mese, nella sessione in cui si punterà a rafforzare il mandato del relatore speciale per i diritti umani in Iran. In Consiglio economico e sociale il 14 dicembre l'Italia ha votato a favore della risoluzione per l'espulsione dell'Iran dalla Commissione sulla condizione delle donne. In maniera compatta con i *partner* dell'Unione europea, l'Italia ha inoltre votato a favore della risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Iran, adottata il 15 dicembre dall'Assemblea generale. Continuiamo a dare messaggi chiari e fermi per esercitare pressioni su Teheran e per ottenere un cambiamento di rotta rispetto alla drammatica fase attuale. Perseguire un confronto, per quanto faticoso, è necessario anche per tutelare la sicurezza e la stabilità della regione, ma non possiamo derogare ai valori su cui si basano la nostra democrazia e la costruzione europea.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, non vi è dubbio che tra il momento in cui abbiamo presentato l'interrogazione e questa giornata sono successe molte cose, molte delle quali fatte dal Governo e credo che sia giusto dare atto della coerenza con cui il Governo, nei vari appuntamenti nazionali e internazionali, si è comportato. Siamo quindi in parte soddisfatti dalla risposta che ci è stata data. Vorremmo però sottolineare come in realtà, nonostante le pressioni dei Paesi più avanzati, delle delle associazioni per i diritti umani e delle agenzie dell'ONU, la repressione in Iran continui a essere molto violenta. Essa assume sempre più delle caratteristiche etniche: penso a quello che succede nelle città curde rispetto a

che sono anche nel nostro Paese e che continuano giustamente a sostenere i loro concittadini che invece manifestano in Iran, di dichiarare i *pasdaran* come organizzazione terroristica. Non mi sfugge che questa scelta, che anche in Europa è molto divisiva, ponga dei problemi, compreso quello che lei stesso, signor

che uccidono nelle strade possano essere sanzionate in quanto organizzazione, non solo in quanto singoli appartenenti a quel corpo.

Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario per la risposta. Noi siamo intervenuti in diverse occasioni su questo tema, ed è intervenuto proprio il ministro Tajani in risposta a un quesito del collega Scalfarotto, quindi non possiamo che prendere

l'indignazione personale e istituzionale del Presidente della Repubblica rispetto a ciò che succede in Iran. Abbiamo sentito delle pressioni e visto i diversi pacchetti sanzionatori che l'Italia si impegna a promuovere anche nelle sedi sovranazionali e internazionali. Abbiamo sentito che il Governo, per bocca del ministro Tajani, ha chiesto all'ambasciatore di non procedere con la repressione e di ascoltare le proteste dei giovani. Purtroppo, signor Sottosegretario, come lei sa bene, queste nostre richieste sono state inascoltate.

di un'intera generazione. Ciò che chiedo al Sottosegretario e a questo Governo è che, oltre alle pressioni internazionali e alle sanzioni economiche, ci sia una continua sensibilizzazione dell'opinione pubblica. pubblica. Non dobbiamo abituarci alla violazione dei diritti umani che avviene in Iran. Questa non è un'ingerenza sulla sovranità di un altro Stato, ma è il modo di adempiere al dovere costituzionale - che noi abbiamo di garantire che la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle giovani generazioni iraniane ci riguarda, perché riguarda tutti i Paesi in cui i diritti e le libertà devono essere rispettati

continuare a chiedere che la repressione in Iran venga fermata. Non solo sono proteste quelle che stanno facendo quei giovani: sono richieste di rispetto dei diritti umani.

con l'interrogazione all'ordine del giorno il senatore Parrini, insieme ad altri senatori, chiede di assumere iniziative al fine di integrare le risorse disponibili per interventi di rigenerazione urbana per l'anno 2022, con l'obiettivo di finanziare tutti i progetti presentati dai Comuni e dichiarati ammissibili. Viene altresì suggerita una modalità di assegnazione delle risorse differente rispetto a quella attualmente praticata, che fa riferimento al criterio dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale, in modo da garantire opportunità di sviluppo su tutto il territorio nazionale. Nel richiamare preliminarmente la cornice legislativa di riferimento, evidenzio che la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, ha previsto specifiche linee di finanziamento per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, dedicate a progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. In particolare, sono stati stanziati 150 milioni di euro per il 2021, 250 per il 2022, 550 milioni per gli anni 2023 e 2024, 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Lo scorso anno l'erogazione dei contributi in questione è stata attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021, a seguito di un'intesa sancita con l'ANCI in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali il 26 novembre del 2020. In quella sede si è convenuto di introdurre, tra i criteri per la selezione dei progetti, quello che fa riferimento all'indice di vulnerabilità sociale e materiale definito dall'Istat, in ragione della necessità di riconoscere una preferenza alle realtà locali più svantaggiate, in coerenza con le finalità dell'intervento legislativo. Rammento anche che, per corrispondere all'esigenza di ampliare la platea dei beneficiari, il legislatore è intervenuto successivamente con il decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17, grazie al quale sono state stanziate ulteriori risorse pari a 905 milioni di euro, che hanno consentito di finanziare tutte le opere che erano state ammesse alla graduatoria finale. Come evidenziato dagli onorevoli interroganti, ulteriori interventi in materia sono stati disposti dalla legge del 30 dicembre 2021, n. 234, che, nell'estendere la categoria dei possibili beneficiari dei contributi, ha previsto per l'anno 2022 l'assegnazione di risorse per progetti di rigenerazione urbana pari a 300 milioni di euro in favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti che, in forma associata, superano detta soglia. La legge appena richiamata prevede che, qualora l'entità delle richieste superi l'ammontare delle risorse, l'attribuzione sia effettuata in favore dei Comuni che presentano un valore più elevato dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale. Con il recente decreto interministeriale del 19 ottobre 2022 sono stati individuati i Comuni beneficiari dei predetti contributi, per un importo complessivo di circa 297 milioni di euro, a fronte di istanze trasmesse da 5.268 enti locali e relative a progetti il cui importo complessivo è risultato ampiamente superiore alle risorse stanziate dalla legge. Pertanto, allo stato attuale risultano presenti in graduatoria ulteriori progetti non finanziati. Assicuro che le criticità segnalate dagli interroganti sono all'attenzione del Governo. In particolare, informo che il Ministero dell'interno, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze e in collaborazione con l'ANCI, ha valutato la possibilità di recuperare risorse da destinare a interventi di rigenerazione urbana. Sono state anche vagliate possibili soluzioni per individuare un correttivo all'utilizzo del criterio dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale, con l'obiettivo di assicurare una più equilibrata distribuzione regionale delle risorse disponibili in relazione alle istanze presentate. Proprio al fine di corrispondere a tali esigenze, con la legge del 13 gennaio 2023, n. 6, in sede di conversione del decreto-legge del 18 novembre 2022, n. 176, è stato introdotto l'articolo 14-*quinquies*, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026. I criteri di riparto del predetto fondo saranno individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna Regione, tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021 n. 234.

Signor Presidente, ovviamente ringrazio il sottosegretario Silli per averci riferito la posizione del Ministero dell'interno circa il problema da me sollevato nell'interrogazione. Non posso tuttavia dichiararmi soddisfatto perché la discriminazione a danno dei Comuni più piccoli, che si è verificata con l'assegnazione delle risorse del PNRR, è pesante. dell'interno del 19 ottobre 2022 lo dicono in maniera inequivocabile; è una discriminazione che ha colpito soprattutto i Comuni sotto i 15.000 abitanti del Centro-Nord del nostro Paese, che sono stati praticamente tenuti fuori da qualsiasi supporto finanziario. Di fronte a un problema così grande, come avrei voluto dire al rappresentante del Ministero dell'interno e dico con garbo al sottosegretario Silli, non basta l'attenzione, serve un'azione

dall'impatto dell'aumento dei prezzi che rischia - lo dico in maniera particolarmente accorata al Governo - di non far partire i cantieri Come sappiamo, l'aumento dei prezzi e il suo impatto sui cantieri è, in proporzione, assai più grande nei Comuni più piccoli perché quelli più grandi qualche spazio di bilancio per assorbire il colpo, anche se è forte per per tutti i Comuni, ce l'hanno. Quelli più piccoli invece questo spazio non ce l'hanno. È perciò necessaria una svolta. Per ora non se ne vedono i segni ed io non posso che approfittare della risposta a questa interrogazione per levare ancora una volta la mia voce affinché si proceda nella direzione giusta.

alle quali risponderanno il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro della salute. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

gli istituti musicali pareggiati e gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), operano nel settore terziario dell'istruzione al pari degli atenei universitari; tali istituzioni si inseriscono nel settore dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), attivano corsi di laurea triennale e magistrale cui si accede con il diploma di scuola secondaria, nonché corsi di specializzazione e dottorati di ricerca, corrispondentemente a quanto avviene negli atenei universitari;

Valutato che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha determinato l'equipollenza dei titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM con quelli universitari; valutato, infine, che per il valore storico, culturale, d'immagine e di eccellenza che tali istituzioni rappresentano per il nostro Paese, un completo adeguamento al settore universitario, analogamente a quanto avvenuto negli Stati membri europei, appare ormai improcrastinabile. Possiamo quindi affermare che, a un sistema di equipollenze "a valle" non è corrisposto uno "a monte", lasciando così irrisolto il problema di come debba essere inquadrato e collocato il personale delle istituzioni AFAM in relazione al personale universitario. Peraltro, ad oggi, la non definitiva equiparazione dei docenti AFAM a quelli universitari ci appare in evidente contrasto con il dettato normativo della legge n. 508 del 1999. A conferma di ciò, basti sottolineare che, a parità di carico orario, un professore delle istituzioni AFAM, a fine carriera, percepisce circa un terzo dello stipendio di un professore universitario. Ciò premesso e considerato, si chiede, quindi, di sapere da lei, signor Ministro, se intenda equiparare a tutti gli effetti le retribuzioni dei docenti AFAM a quelle dei professori universitari, garantendo al sistema AFAM e ai suoi professori una maggiore dignità, in linea con tutti gli altri Paesi dell'Unione europea.

Pirondini e il Gruppo parlamentare a cui appartiene per avere richiamato l'attenzione sull'Alta formazione artistica musicale e coreutica, un settore spesso non sufficientemente valorizzato nel dibattito pubblico, ma che, al contrario, rappresenta un patrimonio prezioso e caratterizzante per il nostro Paese. Sin dall'inizio del mandato che mi onoro di ricoprire al Ministero dell'università e della ricerca, ho considerato l'AFAM come uno dei pilastri delle competenze del Ministero, assolutamente al pari dell'università e della ricerca. Un ulteriore elemento portante del nostro sistema di infrastrutture creative, dal grande valore educativo ma anche dall'enorme potenziale economico; un veicolo culturale ed identitario, capace di intercettare il desiderio diffuso nel mondo di avvicinarsi alla nostra cultura e al nostro capitale umano e di esperienze. Lo dimostra l'altissimo numero di iscritti stranieri ai corsi AFS. Sono circa 13.000 studenti, su un numero complessivo di 83.000, per un tasso pari al 15 per cento del totale, in proporzione ben superiore a quanto avviene nelle università. Il dialogo in Parlamento sulle prospettive del settore è e rimane aperto, come ha dimostrato l'ultima legge di bilancio nella quale, con un emendamento del vostro Gruppo e con il sostegno del Governo, sono stati aumentati i fondi delle istituzioni AFAM per iniziative e servizi a beneficio degli studenti con disabilità. Più in generale, conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) meritano un investimento di fiducia e attenzione all'altezza delle aspettative di un corpo docente di qualità. L'obiettivo è condiviso: applicare compiutamente la riforma avviata ormai nel lontano 1999 e che ancora abbisogna di interventi attuativi che, come ricordava giustamente il collega interrogante Pirondini, solo oggi, dopo un lungo percorso anche attraverso il Consiglio di Stato, sono prossimi a giungere al traguardo. Signora Presidente, sono quasi alla conclusione, ma ci terrei a sottolineare un paio di aspetti. L'intero settore è oggetto di un'ampia rivisitazione che tocca i diversi temi del reclutamento dei docenti, dell'autonomia didattica delle istituzioni e, in prospettiva, anche della loro *governance.* Questa riflessione è stata condotta mediante il doveroso coinvolgimento dei protagonisti e dei rappresentanti del mondo AFAM, che costituiscono una comunità plurale, nella quale è presente un'ampia dialettica sulle prospettive del settore. Gli argomenti di confronto sono stati e sono molteplici e tra questi il livello retributivo costituisce una parte importante del tema complessivo. Bisogna valutare anche l'inquadramento giuridico e contrattuale del personale, rispetto al quale si confrontano posizioni a sostegno del modello costituito dal settore scolastico e altre, come quella rappresentata in questa sede dall'interrogante, rivolte invece al modello del personale docente universitario. È bene ricordare, tuttavia, che ciascuno di questi modelli è caratterizzato da regimi specifici e modalità di selezione e reclutamento diversi, nessuno dei quali è immediatamente applicabile al mondo AFAM senza i dovuti adattamenti. Sarà mio compito ascoltare queste diverse sensibilità e contribuire all'individuazione di una sintesi, che tenga conto delle specificità del mondo AFAM e della pluralità dei suoi orientamenti diffusi tra i suoi docenti e nelle sue istituzioni.

è previsto anche rispetto a quanto ci segnala l'Unione europea. Da questo punto di vista speriamo che possa essere l'inizio di un percorso; non abbiamo la risposta che magari avremmo voluto sentire oggi, ma speriamo si possa andare in una direzione corretta. Per quanto riguarda un lavoro di collaborazione nell'ottica di risolvere questo problema, sappia che il MoVimento 5 Stelle c'è. Signora Presidente, onorevoli colleghi, sottopongo oggi all'attenzione dell'Assemblea e del ministro Schillaci, che ringrazio per la sua disponibilità, un argomento su cui il Governo, fin dall'inizio, ha posto la massima attenzione. Parliamo di salute, di cure e di assistenza ai soggetti più fragili della nostra popolazione, come anziani, persone non autosufficienti, persone con disabilità, malati cronici, bambini. La pandemia che ci siamo lasciati alle spalle ha coniato il termine «fragili»: parliamo di tre milioni di anziani non autosufficienti che, secondo le stime, raddoppieranno entro il 2030, di 6 milioni di persone con disabilità, la cui metà soffre purtroppo di gravi limitazioni che impediscono loro di svolgere attività abituali, ma anche di bambini e malati cronici che richiedono un'assistenza continuativa e costante. Secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità, sei anziani su dieci sono colpiti da una malattia cronica e uno su quattro ne ha due o più. Se diagnosi, assistenza e cure sono necessarie per queste categorie di persone, lo sono ancora di più quando parliamo, ad esempio, di lotta al cancro: il fattore chiave è la prevenzione. A causa della pandemia, nel 2020 sono saltati 2,5 milioni di *screening* oncologici. Siamo tutti ben consapevoli di quanto sia importante una diagnosi precoce quando parliamo, ad esempio, di tumori. Quello che emerge è che sono ancora tanti i ritardi delle Regioni nel recupero delle prestazioni sanitarie rinviate a causa del Covid, nonostante i fondi destinati a tale scopo. Le liste di attesa costituiscono purtroppo una barriera troppo spesso insormontabile per accedere a visite e accertamenti diagnostici: giorni per una mammografia, un anno per TAC ed ecografie, sei mesi per una risonanza. È un problema nazionale, quello delle liste d'attesa, che riguarda purtroppo Regioni virtuose, ma in generale tutte le Regioni italiane. infatti, i centri unici di prenotazione, non riuscendo a rispettare le date indicate nella prescrizione del medico, mettono i pazienti in *standby.* Dunque, le lunghe liste di attesa rischiano seriamente di diventare un muro che impedisce soprattutto ai soggetti più fragili, di cui parlavo all'inizio, di accedere ai servizi sanitari. I canali di accesso ai CUP attraverso i *call center* non riescono ad intercettare la domanda di servizi di tutte quelle persone che, pur bisognose di cure urgenti, non hanno corsie preferenziali di accesso. Chiedo al Ministro quali fondi e quali iniziative siano state approntate per risolvere queste criticità e soprattutto se non ritenga opportuno individuare nuovi percorsi di priorità di accesso alle cure ambulatoriali e ospedaliere e alle diagnosi, in particolar modo per tutelare le fasce per tutelare le fasce sociali più deboli della nostra popolazione: anziani, disabili, persone non autosufficienti, malati cronici e pazienti oncologici. Sommessamente ricordo al Ministro la grave mancanza di medici, che purtroppo è un altro problema che grava su tutti noi.

rammento il decreto del Ministero della salute del 20 agosto 2019, in materia di ripartizione tra le Regioni dei fondi per la riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, che ha consentito l'attivazione di una serie di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni secondo il principio della appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, anche in osservanza delle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste d'attesa. Sebbene le iniziative poste in atto non siano esclusivamente destinate ai soggetti fragili, le stesse hanno favorito una rapida ed avanzata digitalizzazione, potenziando la fruibilità dell'accesso dei pazienti nella direzione di un forte efficientamento dei sistemi di prenotazione. Quanto all'accessibilità delle prestazioni erogate, comunico che l'osservatorio nazionale delle liste d'attesa ha emanato in data 16 gennaio scorso le linee di indirizzo relative ai requisiti e monitoraggio delle sezioni dedicate ai tempi e alle liste di attesa sui siti *web* di Regioni, Province autonome e aziende sanitarie. Dette linee contengono le indicazioni per uniformare e rendere chiare e fruibili ai cittadini le informazioni sui tempi di attesa, sulle modalità di accesso alle cure, nelle quali è stato dato uno specifico risalto agli aspetti di trasparenza, accessibilità e fruibilità per qualunque tipo di utenza. Il monitoraggio è in capo alle Regioni e al Ministero della salute. Tra gli impegni derivanti dal vigente Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, rientrano la definizione e l'applicazione da parte delle Regioni dei percorsi di tutela, ovvero l'attivazione di modalità alternative di accesso alle prestazioni nei casi in cui ai cittadini non possa essere assicurata la prestazione entro i limiti previsti dalle Regioni. Ricordo inoltre che sono già attive in fase di prenotazione le cosiddette classi di priorità, che tengono conto dell'urgenza delle prestazioni per l'accesso alle prestazioni ambulatoriali, così come sono previste nel Piano nazionale di governo delle liste d'attesa le classi di priorità di ricovero, che tengono conto delle specifiche patologie e condizioni in cui versano le persone fragili: i disabili, le persone non autosufficienti, i malati oncologici gravi. Sempre sulle liste d'attesa, ricordo che nel 2022 sono state rese disponibili risorse pari a 500 milioni di euro, di cui 150 milioni per consentire lo smaltimento delle liste d'attesa tramite ricorso alle strutture private accreditate. Tenuto conto che al termine dell'anno 2022 non tutte le risorse erano state utilizzate, per consentire nel corso di quest'anno la prosecuzione delle attività già avviate, mi sono attivato affinché in fase di conversione in legge del decreto-legge n. 198 del 2022 in materia di termini legislativi possa essere approvata la proroga anche per il 2023. Quanto ai servizi di assistenza domiciliare, ricordo che il decreto del Ministero della salute del 23 maggio 2022 ha riformato l'assistenza territoriale e ha definito le cure domiciliari come un servizio a valenza distrettuale, finalizzato all'erogazione a domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità variabile, nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza, introducendo lo *standard* organizzativo del 10 per cento della popolazione *over* sessantacinque anni, da prendere in carico progressivamente, con monitoraggio a cura dell'Agenzia Da ultimo, cito l'intesa in Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre scorso, che ha ripartito le risorse per l'assistenza domiciliare, di cui all'investimento componente 1 - missione 6 del Piano

migliori per dare risposte ai cittadini, soprattutto a quelli che hanno più bisogno. Credo che questo sia uno degli aspetti prioritari di uno Stato: senza la salute non ci può essere null'altro e credo che questo sia l'aspetto primario. Proprio per questo motivo e per il percorso a cui ha appena Grazie

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, sono qui a parlarvi dell'ospedale di Malcesine, sul lago di Garda, in provincia di Verona, che il 29 marzo del 2007 è stato riconosciuto Centro di riferimento nazionale per lo studio e la cura degli esiti tardivi della poliomielite dalla Conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. L'Italia è stata ufficialmente certificata *polio-free* il 21 giugno 2002. Essa è ricomparsa ultimamente in alcuni Paesi, in altri non è ancora stata debellata e va continuamente monitorata per impedire la sua reintroduzione nel nostro Paese. Inoltre, si stima che in Italia oltre 70.000 persone, sopravvissute alla malattia, ne patiscono tuttora gli esiti. Nel corso dei decenni, l'ospedale di Malcesine, sul lago di Garda, è stato l'unico a non cessare mai l'attività a favore dei pazienti polio, mantenendo sempre dei letti a loro dedicati, tenendo viva la conoscenza e l'esperienza maturata dall'applicazione di tecniche e trattamenti effettuati su questo tipo di malattia. Il 30 novembre 2014, presso la Camera dei deputati, l'ordine del giorno 249 alla legge di stabilità per il 2015 ha impegnato il Governo a valutare l'opportunità di farsi promotore di un accordo affinché tutte le Regioni e le Province autonome concorrano con fondi alla gestione del centro nazionale

provocando la comprensibile preoccupazione da parte dei pazienti che provengono da tutte le regioni d'Italia, delle loro famiglie e dal personale medico. Forte preoccupazione condivisa anche dalla popolazione tra Malcesine e Lazise, che si trova in forte difficoltà rispetto alla copertura sanitaria, con milioni di presenze di turisti che ogni anno visitano la sponda veronese del lago di Garda e ai quali, l'ospedale di Malcesine, attualmente garantisce un punto di primo intervento; Oggi la struttura è parzialmente operante. Secondo una ricognizione effettuata da FP CGIL Verona e dall'Associazione interregionale disabili motori (AIDM), con sede interna all'ospedale, mancano più della metà degli 80 posti letto previsti dal piano socio-sanitario della Regione Veneto, con più o meno 800 disabili in lista di attesa che

Presidente, senatrice Aurora Floridia, con riferimento al quesito in esame ricordo che il Centro nazionale per esiti tardivi della poliomielite anteriore acuta dell'ospedale di Malcesine accoglie pazienti da tutte le Regioni d'Italia. L'ospedale in questione è inquadrato quale punto di primo intervento con attività H24 e numero di accessi da 3.000 a 6.000. Nella programmazione ospedaliera il citato ospedale è inquadrato come struttura riabilitativa *post* acuzie, con 50 posti letto di codice 56 programmati. La trasformazione verso il sistema 118, e quindi in postazione territoriale per emergenza, prevista dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, è stata differita in considerazione non solo dell'elevato afflusso turistico nella zona, ma anche per la distanza dal più vicino pronto soccorso, raggiungibile peraltro solo tramite una viabilità difficoltosa. Come riferiscono la Regione Veneto e l'azienda ULSS 9 Scaligera di Verona, le modalità di accoglimento dei pazienti sono state recentemente riviste a favore di un progressivo azzeramento del tempo medio di attesa per il ricovero. Nel corso del 2022 sono state prese in carico le richieste pervenute con con di fatto il loro azzeramento programmato entro i primi mesi del 2023, e a partire dal primo aprile 2023 in poi sarà attiva un'agenda di prenotazione con una nuova modalità di accesso, basata su criteri di priorità clinica valutati dallo specialista fisiatra prima dell'inserimento nella stessa. I posti letto attualmente attivi sono 29, tutti in un unico piano. Al fine di portare a compimento la programmazione prevista dalle schede regionali, *ex* deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 2019, è necessario un ulteriore incremento di organico nella dirigenza medica e delle professioni sanitarie, e operatori sociosanitari, per il cui reclutamento sono attivate varie procedure concorsuali, non sempre però pari a quello desiderato, anche probabilmente in ragione della posizione decentrata della struttura, non attrattiva per le risorse acquisibili in questo particolare scenario della sanità nazionale. L'azienda ULSS 9 ha sempre espresso particolare sensibilità per le cure altamente specialistiche in favore dei pazienti con esiti tardivi da poliomielite, tanto che il servizio di degenza non è stato mai interrotto, nemmeno durante le fasi di maggiore pressione della pandemia da Covid-19 sui servizi sanitari. È volontà dell'azienda ULSS 9, condivisa dalla Regione Veneto e dal Dicastero di cui ho la responsabilità, di portare al pieno funzionamento il Centro nazionale per gli esiti tardivi della poliomielite di Malcesine non appena si potrà completare la dotazione di organico, come previsto dalla normativa. In data 23 febbraio sarà espletata la prova di selezione del direttore di struttura complessa di riabilitazione. I lavori effettuati presso il presidio ospedaliero sono sempre stati condivisi con l'associazione AIDM (Associazione interregionale disabili Concludo dicendo che condividerò tutte le iniziative e azioni possibili, ive incluse quelle per garantire le necessarie risorse finanziarie, per dare sempre un'ampia e tempestiva risposta ai bisogni di salute dei cittadini che presentano esiti tardivi di poliomielite e che trovano nel nosocomio di Malcesine un centro di eccellenza per la loro cura.

L'ha detto anche lei: degli 80 posti letto riservati dalle schede ospedaliere al momento lei ne ha citati 29, a me ne risultano 25, comunque quelli sono. C'è quindi una difficoltà oggettiva, per cui accolgo con favore la sua

che, oltre ad aver avuto la sfortuna di avere contratto questa terribile malattia da anni, sentono un forte disinteresse da parte del Servizio sanitario regionale e anche nazionale. Noi, lo Stato, abbiamo in mano un gioiello che, che, per scelte politiche effettuate in passato, è stato riposto in cantina e adesso merita di tornare quello che era. Si potrebbero veramente cogliere e sfruttare diverse funzioni di questo ospedale che, essendo in una posizione invidiabile, proprio sulle rive del lago

finestra") *(Az-IV-RE)*. Signor Ministro, la carenza di personale sanitario - come sappiamo - può stimarsi attorno ai 25.000 medici e ai 63.000 infermieri, a fronte di un sistema sanitario che, in ragione anche della

sono stimati in circa 21.000 unità per gli infermieri e in quasi 30.000 unità per i medici. Oltre a questa cronica carenza di personale, destinata ad aggravarsi ulteriormente dopo la pandemia, sappiamo che non si potranno offrire risposte in tempi rapidi a tutti i pazienti, dal punto di vista sia delle liste d'attesa, sia dei fenomeni sanitari e sociali della rinuncia alle Secondo il *report* dell'osservatorio GIMBE, la riduzione complessiva delle prestazioni sanitarie si attesta su un valore di meno 144,5 milioni, di cui la maggior parte in strutture pubbliche, con una diminuzione media del 40 per cento delle attività di *screening* per condizioni cliniche il cui esito è fortemente condizionato dalla tempestività della diagnosi (pensiamo solo alle mammografie, per fare un esempio). I tempi di attesa mediamente superano l'anno e spesso riguardano non solo le tempistiche relative alla diagnosi, ma anche quelle di interventi terapeutici e assistenziali-riabilitativi, che finiscono inesorabilmente per aggravare il quadro clinico del paziente. Secondo il rapporto civico sulla salute di Cittadinanzattiva, almeno l'11 per cento delle persone ha già rinunciato a visite e a esami diagnostici specialistici, anche per problemi economici o legati alle difficoltà di accesso al servizio, con Regioni C'è un problema quindi, Ministro, che lei conosce bene, di prevenzione che viene meno, di strutture sanitarie che, nonostante le risorse stanziate nel corso della pandemia, hanno anche bisogno, per il 70 per cento, di urgenti interventi di rinnovamento. Per non pensare a quello che è accaduto, anche dal punto di vista drammatico, al Pertini di Roma lo scorso gennaio. Concludo dicendo, Ministro, che c'è anche una carenza di alcuni farmaci - come lei sa bene - dagli antibiotici agli antipiretici, persino agli antitumorali. Con questo *question time* vorremmo sapere qual è la sua linea e quali saranno le sue iniziative per far fronte a queste grandi e importanti criticità, perché

in particolare dei vincoli assunzionali, ha determinato da anni una significativa riduzione del personale del Servizio sanitario nazionale. Andiamo per gradi, esaminando le criticità sollevate. Sul tema del finanziamento del Sistema sanitario nazionale, tengo a ribadire quanto già comunicato in fase di replica delle mie linee programmatiche e cioè che, dopo un periodo di definanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, che addirittura negli anni dal 2012 al 2019 ha visto incrementi annui in valore percentuale negativo, la legge di bilancio per il 2023 ha previsto un incremento del Fondo sanitario nazionale. In particolare, il comma 535 ha disposto che il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*

Per l'anno 2023, una gran quota dell'incremento per il primo periodo, pari a 1,4 miliardi di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Tornando al personale sanitario, con riferimento al decennio 2009-2019, il personale dipendente a tempo indeterminato del comparto sanità è diminuito complessivamente del 6,5 passando da 693.600 unità del 31 dicembre 2009 a 648.547 del 31 dicembre 2019. Per quanto riguarda il solo personale del ruolo sanitario comparto dirigenza, la diminuzione registrata nel decennio 2009-2019

a 107.044 unità. Per quanto concerne invece il personale infermieristico, il decremento di dipendenti a tempo indeterminato registrato nel medesimo periodo è stato pari a meno 3 Questa contrazione di risorse ha finito per generare nel medio periodo una grave carenza di professionisti sanitari nelle strutture con riferimento soprattutto ad alcuni settori. Questo ha comportato difficoltà nell'organizzazione e nella gestione dei servizi sanitari. La situazione emergenziale ha ulteriormente acuito le difficoltà del sistema sin dal manifestarsi della pandemia da Covid-19. Questo ha reso necessario adottare misure straordinarie per consentire alle Regioni di poter reclutare in tempi rapidissimi i professionisti, stanziando all'uopo le risorse necessarie. Anche per effetto di queste misure, i dati del conto annuale a partire dal 2020 mostrano un'inversione di *trend* decrescente registrato fino al 2019. Nel 2020 il personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato del comparto sanità è cresciuto del 2,3 per cento rispetto all'anno precedente. Proprio nella consapevolezza delle criticità connesse alla carenza del personale sanitario, ho proceduto intanto prorogando le misure straordinarie già vigenti non solo nella legge di bilancio per il 2023, ma anche mediante le disposizioni del decreto legislativo proroga termini, in ordine al quale la legge di conversione sarà integrata con ulteriori proroghe delle misure che consentono alle strutture del Sistema sanitario nazionale di fronteggiare l'emergenza del personale. Ci tengo a precisare che la mia strategia di azione non si esaurisce solo prorogando misure emergenziali. Per rimediare agli errori del passato ribadisco il mio impegno a trovare le risorse necessarie per superare il blocco del *turnover*, ma soprattutto a mettere in campo una strategia generale che riveda l'intero assetto relativo al reclutamento del personale sanitario con misure di carattere sistemico, anche intervenendo d'intesa con il Ministro dell'università sul tema degli accessi ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione. Quanto alla necessità di valorizzare la professionalità acquisita dal personale sanitario che ha prestato servizio durante l'emergenza pandemica, ricordo che l'articolo 1, comma 268, lettera *b)*, della legge di bilancio per il 2022 ha previsto la possibilità per gli enti del Sistema sanitario nazionale di stabilizzare il personale assunto a tempo determinato che abbia svolto un periodo rilevante del proprio servizio nel corso dell'emergenza pandemica. Al fine di ampliare l'ambito di applicazione della stessa, l'articolo 1, comma 528, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha esteso fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di ricorrere alle predette procedure. Con specifico riferimento al tema delle strutture, è mia intenzione rivedere il decreto ministeriale n. 70 del 2015, che ha disciplinato gli *standard* delle strutture ospedaliere, per adeguare i contenuti alla domanda di assistenza. In ordine alle liste di attesa per i tempi contingentati a disposizione, rinvio a quanto riferito al senatore De Poli. Mi limito a ribadire il mio impegno a prorogare le misure esistenti, che già prevedono i piani regionali. Sul tema della carenza farmaci, infine, a gennaio scorso ho convocato il tavolo di lavoro permanente sull'approvvigionamento per definire la reale entità del fenomeno e indicare proposte risolutive, alla presenza dei rappresentanti del Ministero della salute, di Aifa, della filiera farmaceutica produttiva, ma soprattutto dei medici di medicina generale. infatti che una misura di contrasto della carenza in esame sia rappresentata dal limitato ricorso alla prescrizione e all'utilizzo dei farmaci equivalenti.

un'analisi più puntuale anche rispetto ad alcune posizioni politiche che non ci convincono.

hanno aumentato la loro aspettativa di vita (e oltre i sessantacinque anni la spesa sanitaria è chiaramente maggiore); abbiamo subito un contraccolpo forte durante l'emergenza Covid, per cui è necessario avere un piano rivoluzionario sulla sanità,

di acquisire i soldi del MES e di immettere 37 miliardi di risorse per poter modernizzare gli apparati diagnostici e i pronto soccorso, al fine di dare una risposta seria alla medicina territoriale. modo, le dico con grande franchezza che mi aspetto che lei sappia intervenire puntualmente sulla scelta sbagliata di continuare a diversificare la sanità da Regione a Regione. Quando parliamo di autonomia dobbiamo estrapolare il tema della sanità e renderla una delle questioni riguardanti l'intero Paese, con una visione unitaria. È da qui, che si può passare per sconfiggere, per esempio, una delle altre grandi piaghe che lei ha citato, e cioè le liste d'attesa. Abbiamo bisogno di progetti che sappiano rivoluzionare anche un po' l'impostazione finora utilizzata. Lo dico perché non c'è nulla di più odioso

criticando il suo ragionamento e considerandolo deludente nella fase attuale, ma anche auspicando che la sua libertà possa portarla a scelte più coraggiose e più giuste nel prossimo futuro.

Ministro, il presidio ospedaliero Agostino Maresca di Torre del Greco, in provincia di Napoli, è stato strutturato fino alla potenzialità di circa 250 posti letti per pazienti acuti, con alti livelli di specializzazione. Al presidio ospedaliero Maresca ricorrono, in caso di emergenza, i cittadini di Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio, ed è accorpato al presidio ospedaliero di Boscotrecase, che serve Boscotrecase, Boscoreale, Trecase e Torre Annunziata; insieme costituiscono gli Ospedali riuniti area vesuviana, con la disponibilità di circa 100 posti letto per acuti, con un bacino totale di utenza di circa 340.000 unità. Il servizio sanitario di assistenza ospedaliera sul territorio di competenza della ASL Napoli 3 Sud risulta inefficace, inefficiente e inappropriato per errata impostazione del piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del decreto ministeriale n. 70 del 2015 decreto del commissario *ad acta* n. 103 del 2018; risultano poi una notevole riduzione dei posti letto per acuti, con conseguente errata classificazione e con dimensionamento del presidio ospedaliero Maresca e degli altri presidi dell'ASL Napoli 3 Sud, un errato conteggio dei posti letto per acuti nella macro area più popolosa della stessa area Napoli 3. I dati evidenziano l'assoluta insufficienza dell'offerta sanitaria sul territorio (0,34 posti letto pubblici per acuti ogni 1.000 abitanti), molto lontana dai parametri previsti dal decreto del commissario n. 49 del 2010 (2,7 posti letto per 1.000 abitanti) e anche dal decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 per il contenimento della spesa sanitaria posti letto per acuti ogni 1.000 abitanti e tasso di ospedalizzazione di 160). Si chiarisce poi che gli indici che recano 2,7 posti letto e 3 posti letto per acuto ogni 1.000 abitanti sono riferiti a strutture pubbliche e private, purché accreditate per il servizio di assistenza ospedaliera secondo il fabbisogno dell'ASL. Tutta la rete ospedaliera di emergenza all'ASL Napoli 3 è strutturalmente insufficiente per assicurare i minimi LEA, e le strutture private accreditate contribuiscono effettivamente alla rete dell'emergenza solo se dotate di adeguato pronto soccorso. Gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e, nell'ambito delle proprie competenze, come voglia intervenire affinché la Regione Campania possa garantire una corretta programmazione, assicurando a tutti i cittadini un servizio di assistenza ospedaliera efficace, efficiente e appropriato, come previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 e come richiesto all'articolo 32 della Costituzione; nonché come intenda salvaguardare l'ospedale Agostino Maresca di Torre del Greco, a tutela della salute dei cittadini, con il potenziamento di ambulatori, reparti e servizi del pronto soccorso di eccellenza per l'intero territorio, ridando dignità ai pazienti e al personale sanitario.

realizzata in conformità al decreto ministeriale n. 70 del 2015. Ha comunicato inoltre che l'ospedale Agostino Maresca di Torre del Greco, sede di pronto soccorso, ha un totale di 150 posti letto programmati e 103 posti letto attivi, di cui 32 Covid. In particolare, i posti letto programmati per il presidio ospedaliero di Torre del Greco sono 150, quelli del presidio ospedaliero di Boscoreale sono 153, i posti letto per acuti sono complessivamente 239. La Regione Campania, in data 28 dicembre 2018, con delibera n. 103, ha approvato il documento recante il piano regionale di programmazione della rete ospedaliera, ai sensi del decreto ministeriale n. 70 del 2015, articolata su macro aree territoriali; macroarea delle Province di Avellino e Benevento, macroarea della Provincia di Caserta, area della Provincia di Napoli con la macroarea della ASL Napoli 1 Centro, la macroarea dell'ASL Napoli 2 Nord, la macroarea dell'ASL Napoli 3 Sud e, infine, la macroarea della Provincia di Salerno. Nel menzionato documento programmatorio la Regione Campania fa presente che, nell'area di Napoli, il patrimonio edilizio della ASL Napoli 3 fa rilevare una carenza di strutture di rilevanti dimensioni, utilizzabili nell'area dell'emergenza urgenza. Ulteriore complessità è rappresentata dalle forti criticità di viabilità esistenti in penisola sorrentina, dove insiste anche un rilevante flusso turistico. Con l'attuazione degli interventi del primo stralcio del programma di edilizia sanitaria si prevede la messa a norma del presidio ospedaliero di Nola, del presidio ospedaliero di Boscoreale-Boscotrecase e del presidio ospedaliero di Torre del Greco, con incremento relativo di posti letto rispetto a quelli attualmente disponibili. Lo *standard* dei posti letto della rete ospedaliera della Regione Campania si compone dell'offerta pubblica e privata accreditata. Nel complesso la media regionale è di 3,4 posti letto per mille abitanti; la media aziendale dell'ASL Napoli 3 Sud tuttavia è pari a 2,2 posti letto per mille abitanti, di cui 1,7 posti letto per acuti e 0,5 posti letto per post-acuti. La Regione segnala che in effetti l'attivazione dei posti letto assegnati viene condizionata dalla carenza del personale sociosanitario. In merito alla necessità di una fattiva collaborazione con le case di cura private, la Regione precisa che sono attivi rapporti contrattuali ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, con 12 case di cura accreditate, le quali operano nel rispetto del tetto di spesa imposto dal decreto legislativo n. 95 del 2012. Per quanto riguarda i profili di competenza del Ministero della salute, rassicuro i senatori che hanno sollevato la questione che sarà garantita, da parte della competente direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero, tutta l'attività istituzionale per verificare che siano rispettati i parametri che consentono un servizio di assistenza ospedaliera efficiente e appropriata nella Regione Campania.

dalla madre. Tale triste accadimento ha portato direttamente alla memoria di molte donne quello che è successo durante il parto. Vi posso portare anche la mia testimonianza: tre parti naturali, tre parti differenti. Dopo trenta ore di travaglio, col secondo, ero veramente esausta. Ho quindi allattato il bambino e, alla sera, ho chiesto alle infermiere, avendo scelto il *rooming

Quindi, io potevo essere nella stessa condizione di quella madre. Voglio portare in quest'Aula, perciò, la voce di tante donne, tante future mamme e neo mamme che magari hanno subìto una violenza ostetrica, anche solo psicologica o verbale, e attenzionare il Governo. La pratica del *rooming

La questione sollevata nel *question time* ha generato, nei giorni scorsi, oltre che una profonda tristezza in tutti noi, anche segnali di allarme per tutte le istituzioni coinvolte. Come noto, il modello *rooming in* consiste nel mantenere il neonato nella stanza della madre H24. Come inteso dalla dichiarazione congiunta OMS ed Unicef, quale elemento fondamentale all'interno di un modello virtuoso organizzativo di percorso nascita, esso è finalizzato alla promozione dell'allattamento materno, al benessere neonatale e allo sviluppo delle competenze genitoriali di entrambi i componenti la coppia. Il *rooming in* offre i vantaggi: facilitazione dello sviluppo delle competenze materne nella cura del proprio bambino, promozione dell'attaccamento e della relazione mamma bambino, processo di *bonding*, riduzione del rischio di infezioni ospedaliere per il neonato, promozione dell'*empowerment* della mamma, dimissione protetta attraverso un'assistenza mirata allo sviluppo della *compliance* materna e facilitazione e sostegno all'avvio e al mantenimento dell'allattamento materno a richiesta del neonato. Il *rooming in* prevede il periodico controllo del benessere materno e neonatale da parte del personale di degenza ostetrica e del nido, il quale deve essere però quantitativamente adeguato alle esigenze assistenziali. Svolte queste considerazioni di carattere generale, tornando al terribile episodio del neonato deceduto all'ospedale Pertini di Roma nella notte fra il 7 e l'8 gennaio scorso, ho dato disposizione alla competente Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero di chiedere una relazione alla Regione Lazio in merito all'evento. Ha avuto luogo anche un'ispezione dei carabinieri del Nas, svolta compatibilmente con le indagini penali della procura in corso. Ho tempestivamente predisposto la convocazione di un gruppo di lavoro di esperti in materia, che stilerà un protocollo di buona pratica clinica per la gestione del modello del *rooming in*, anche in termini di fabbisogno del personale e anche per la valutazione dei casi in cui si possa derogare a questo modello nell'interesse esclusivo delle neomamme e dei neonati.

come risposta anche per invertire la tendenza al cosiddetto inverno demografico. È sicuramente una rassicurazione importante per le donne e le future mamme sapere che il Governo voglia aiutarle in un percorso di fertilità, procreazione, assistenza preparto con corsi di preparazione alla maternità e al parto, attenzione durante e dopo il parto, con la pratica del *rooming in*, come diceva il signor Ministro, affiancate dal *partner* e dai familiari, che deve essere però uniforme tra le Regioni e gli ospedali, senza avere alcun tipo di differenza. L'assistenza all'allattamento e *post* parto sono tematiche legate all'alfabetizzazione sanitaria, che è importante per le future mamme e i futuri papà. intervento ringraziandola, perché sicuramente ci deve essere la libertà di fare dei figli ed è questo il messaggio che dobbiamo dare: fare figli è nella nostra natura e deve essere bello poterlo fare insieme, sapendo che il Governo è al nostro fianco. Ed è una libertà di crescita personale, familiare e sociale.

Tre anni fa ho preso servizio presso l'università di Padova come direttore dell'unità complessa di microbiologia e microbiologia clinica e direttore della scuola di specializzazione e con grande sorpresa ho appreso che gli studenti specializzandi laureati in biologia, contrariamente ai colleghi medici, non usufruivano di nessuna borsa di studio, nonostante avessero gli stessi obblighi formativi e assistenziali. Questa odiosa e iniqua disparità di trattamento interessa anche gli studenti che attengono le scuole di specializzazione riservate alle categorie di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, che contribuiscono al funzionamento del nostro Servizio sanitario nazionale, nonostante il loro percorso universitario sia equiparato per legge agli specializzandi laureati in medicina. Infatti, il decreto interministeriale n. 710 del 2016, di riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici, ha formalmente uniformato i percorsi formativi tra le due figure. Pertanto, indipendentemente dalla laurea, è previsto che il 70 per cento formativi maturi attraverso tirocini e pratiche, lavorando quindi nei nostri ospedali almeno 34 ore a settimana. Questi specializzandi che non beneficiano della borsa di studio sono più di 1.500. Colleghi, noi chiediamo a queste persone di lavorare ogni settimana *gratis* per il funzionamento del nostro Sistema sanitario nazionale. La pandemia ha reso ancora più odiosa questa situazione. Ricordo a tutti quanti noi, che sono stati i nostri specializzandi ad aver analizzato ogni giorno centinaia di migliaia di tamponi, i nostri specializzandi farmacisti ad avere assicurato i dispositivi di protezione e i medicinali, i nostri fisici ad avere assicurato il corretto funzionamento dei macchinari. Questo solo per fare alcuni esempi. Il decreto-legge rilancio ha stanziato 95 milioni per finanziare 4.200 contratti di specializzazione in più, ma purtroppo nessuna di queste risorse è destinata ai non medici. Signor Ministro, lei non è responsabile di questa situazione, ma, a differenza dei suoi predecessori, lei è un medico, ha lavorato a lungo in ospedale, è rettore di una importante università, quindi non può esserle sfuggita questa disparità di trattamento che non trova senso né giustificazione, che l'Italia sta sfruttando il lavoro di giovani. Per questo le chiedo di sapere quali iniziative lei intenda adottare nell'ambito delle sue competenze al fine di superare questa assurda disparità di trattamento e quali risorse intende reperire. PRESIDENTE.

da parte dei Governi che ci hanno preceduto. Probabilmente, come spesso accade in vicende analoghe, la causa è da ritrovarsi nella mancanza di adeguate coperture finanziarie. Aggiungo che il tema investe per competenza anche il Ministero dell'università, per cui saremo affiancati sulle iniziative da assumere. Inoltre, proprio per evidenziare quanto la criticità sia risalente, comunico che sin dal 2015 si è instaurato un significativo filone di contenzioso. Ciò premesso, passo ad affrontare nel merito la questione posta, ricordando che la corresponsione della cosiddetta adeguata remunerazione agli specializzandi medici discende dalle direttive comunitarie 82/76/CEE, 93/16/CEE e 2500/36 CEE, che hanno previsto l'obbligo per gli Stati membri di corrispondere un giusto compenso in favore dei soli medici durante la formazione specialistica, quindi le direttive risalgono rispettivamente al 1982 e al 2005, mentre un simile obbligo comunitario non è stato purtroppo previsto anche per le altre figure professionali quali veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici. La legge n. 401 del 2000 richiamata nel quesito, pur prevedendo l'articolo 8, comma 1, che il numero dei laureati non medici iscrivibili alle scuole di specializzazioni *post* laurea è determinato secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, non ha tuttavia individuato una congrua copertura economica. Infatti, ai sensi della predetta predisposizione, resta ferma la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste. Atteso il mancato stanziamento di risorse aggiuntive, l'applicabilità della citata disposizione ha presentato profili di criticità che hanno indotto il legislatore, nelle more di una definizione organica della materia e per evitare un arresto nella formazione specialistica dei predetti professionisti sanitari, a prevedere con l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito dalla legge n. 89 del 2016, l'attivazione delle scuole di specializzazione non mediche in deroga al predetto articolo 8, comma 1 della legge n. 401 del 2000. Va peraltro evidenziato che ai sensi del decreto interministeriale del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della salute del 16 settembre 2016, recante riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici, le differenze riguardano non solo il trattamento economico dei professionisti sanitari iscritti alle relative scuole, ma anche ulteriori aspetti, quali le modalità di selezione per l'accesso, le modalità di accreditamento delle scuole di specializzazione delle strutture facenti parte della rete formativa delle scuole stesse. In tal senso, una piena equiparazione dei diversi professionisti non può prescindere da un intervento normativo di più ampio respiro che preveda il necessario coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della individuazione delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dal finanziamento dei contratti di specializzazione da assegnare anche ai predetti professionisti. Da ultimo, rappresento che nell'ambito dei lavori dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica istituto presso il Ministero dell'università e della ricerca, cui il Ministero della salute partecipa con propri rappresentanti, è stato attivato un gruppo di lavoro per l'approfondimento delle questioni relative alle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica anche ai fini della definizione dei requisiti per l'accreditamento.

che non ci obbliga, di fatto sfruttiamo il lavoro di migliaia di studenti senza pagarli creando una situazione intollerabile che poi si ripercuote anche sul funzionamento delle scuole stesse di specializzazione. Prendo atto della sua buona volontà e anche di quella del Ministro dell'università e della ricerca. Ci faremo carico di presentare un disegno di legge che spero venga condiviso da tutti e conto su di lei perché possa trovare le risorse per la piena applicazione di questa iniziativa e per mettere fine a questa situazione iniqua. *(Applausi)*.

Ministro, il 4 febbraio ricorre la 23ª Giornata mondiale contro il cancro. I numeri forniti dall'Associazione italiana di oncologia, nel rapporto intitolato «I numeri del cancro in Italia 2022», stimano

evidente che sulle stime pesano i gravi ritardi accumulati durante la pandemia da Covid-19, specialmente nelle prestazioni diagnostiche e di *follow-up* previste dai modelli di cura e dai piani terapeutici. Il Piano oncologico nazionale: documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione del contrasto del cancro 2023-2027, adottato il 26 gennaio 2023, con l'intesa in Conferenza Stato-Regioni, ha lo scopo di migliorare il percorso complessivo di lotta alle patologie neoplastiche, in termini di efficacia, efficienza, appropriatezza e gradimento dei pazienti, con una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico e con il grande obiettivo della riduzione, fino all'eliminazione, delle disuguaglianze nell'accesso agli interventi di prevenzione e cura, ad esempio nel campo della genomica dei tumori, per una prevenzione e una terapia sempre più personalizzate, da rendere disponibili da parte degli organi dello Stato. la interrogo dunque per sapere quali sono le azioni che intende intraprendere, rispettando ogni singola voce indicata nel piano, per rafforzare la prevenzione, incrementare la diagnosi precoce, migliorare l'accesso alle terapie e garantire, anche a tutti coloro che hanno superato la fase acuta della malattia, i servizi sanitari e sociali di cui continuano ad avere bisogno.

sia come medico che come Ministro della salute, tanto che la prevenzione e la cura del cancro sono in cima alle priorità del nostro Dicastero. Il Piano oncologico nazionale, documento di pianificazione e indirizzo per la prevenzione del contrasto del cancro 2023-2027, dopo un lungo *iter*, è stato approvato mediante intesa in sede di Conferenza Stato Regioni lo scorso 26 gennaio. La priorità del Ministero della salute è una priorità non solo nazionale e infatti il 4 febbraio 2023

Europe's beating cancer plan - nel senso che individua obiettivi e linee strategiche corredate da alcuni indicatori di monitoraggio, allo scopo di migliorare il percorso complessivo di lotta alle patologie neoplastiche in termini di efficacia, efficienza, appropriatezza, *empowerment*, gradimento dei pazienti e a contenere i costi sanitari e sociali da essi determinate. Per il suo finanziamento, per gli anni 2023 e 2024, guardo con particolare favore all'emendamento inserito disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, teso ad istituire, nello stato di previsione del Ministero della salute, un apposito fondo, denominato Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027. Tale fondo, che nasce con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni, è destinato al potenziamento delle strategie e delle azioni per prevenzione, diagnosi, cura e assistenza del malato oncologico, definite nel piano oncologico nazionale. Le potenzialità di detto piano sono rappresentate da un approccio globale intersettoriale, con una maggiore integrazione tra prevenzione, diagnosi precoce e presa in carico, compreso il miglioramento delle cure e la prevenzione delle recidive, ponendo l'attenzione sulla centralità del malato e sulla riduzione o eliminazione delle diseguaglianze nell'accesso agli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione. Ai fini dell'ottimizzazione del percorso terapeutico sarà fondamentale la piena realizzazione, in tutte le Regioni, delle reti oncologiche, nell'ottica di favorire un'assistenza sempre più domiciliare e integrata tra ospedale e servizi territoriali, avvalendosi anche delle case di comunità, tramite l'implementazione della telemedicina e la valorizzazione del ruolo di medici di famiglia, pediatri e infermieri di comunità. In continuità con il tema del percorso, viene affrontato quello della riabilitazione del malato oncologico. Infatti, la guarigione, intesa come completo recupero fisico, psichico e sociale, il raggiungimento dell'autonomia relazionale e il reinserimento occupazionale dei pazienti guariti o dei pazienti cronicizzati costituiscono obiettivi non solo di politica sanitaria, ma di *welfare* in generale. Ciò consentirà anche di evitare inutili e gravosi spostamenti del malato, permetterà di assicurare una presa in carico precoce e globale per ogni paziente, già in fase di fondato sospetto. Altro obiettivo importante è mantenere lo stato di benessere raggiunto, prevenire l'insorgenza di patologie cronico-degenerative e la ripresa della malattia. Sono fiducioso che le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle competenze istituzionali, provvederanno a recepire il documento nell'ambito dei territori di competenza con provvedimenti regionali, individuando le soluzioni organizzative più idonee per garantire cure e percorsi di riabilitazione appropriati ed uguali su tutto il territorio nazionale. il ministro, professor Schillaci. Ho la netta consapevolezza della sua attenzione verso questa problematica, veramente centrale centrale nell'attuale emergenza rappresentata dal *post* pandemia. L'enorme mole di prestazioni sospese, che va ad accrescere le già già insopportabili liste d'attesa datate da prima del 2019, impongono una sorta di piano Marshall sulle terapie oncologiche. Avverto una grande sensibilità da parte sua rispetto all'equità nella distribuzione delle prestazioni sanitarie oncologiche, che deve interrompere quella transumanza di pazienti dal Sud verso il Nord, questa differenza nella distribuzione dei LEA, che è cosa veramente da Paese poco civile, e soprattutto consentire la reale presa in carico di questi pazienti, che sono di fatto pazienti fragili. Questa presa in carico non può non tener conto anche della fase di *post* acuzie in cui si trova il malato oncologico, che deve continuare per lunghi anni ad effettuare i cosiddetti *follow-up* e sotto una sorta di spada di Damocle, rispetto alla quale ha bisogno di sentire vicino lo Stato, ha bisogno di essere assistito e preso effettivamente in carico anche dal punto di vista psicologico. So, Ministro, di trovare in lei una persona di grande sensibilità e su questo facciamo affidamento anche nel lavoro parlamentare che ci vedrà impegnati nel prossimo provvedimento di proroga termini con un emendamento a firma di Fratelli d'Italia che prevede, appunto, il finanziamento del biennio di questo Piano oncologico nazionale. *(Applausi)*.

*(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi giorni il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara ha riferito che gli stipendi dei professori potrebbero subire una differenziazione regionale. Questa dichiarazione, però, non ci lascia sbigottiti, perché è la riconferma che questo Governo sta lavorando solamente per una parte del Paese, mettendo a serio rischio la tenuta dell'unità nazionale, un'unità ostaggio di provvedimenti pericolosi, dall'autonomia differenziata alle gabbie salariali. Non come senatrice, ma da ex insegnante, ritengo che parametrare gli stipendi in base al luogo di residenza frammenterebbe ulteriormente l'Italia, dividendo il corpo docenti in lavoratori di serie A e di serie B. Un principio di *apartheid* che mi ricorda quella vecchia proposta del ministro Matteo Salvini, che suggerì di destinare alcune carrozze della metropolitana di Milano ai soli milanesi. Sia chiaro: condivido la necessità di aumentare gli stipendi agli insegnanti, purché ciò avvenga da Trieste a Lampedusa. Perciò è sbagliato, oltre che propagandistico, sostenere che questa misura debba essere estesa solo in quei territori in cui il costo della vita è maggiore, significherebbe ignorare la sperequazione economica a cui è da sempre soggetto il Meridione, che solo dal 2000 al 2017 si è visto sottrarre 840 miliardi di euro, stando a un recente *report* di Eurispes. Vorrebbe dire ignorare che il Sud sia l'area più povera d'Europa, secondo un rapporto di Eurostat. Vorrebbe dire ignorare che nelle Regioni meridionali, in assenza di quei sussidi che ora la maggioranza vuole tagliare, l'incidenza della povertà assoluta fra le famiglie avrebbe raggiunto il picco del 13 per cento, secondo lo Svimez. Vorrebbe dire ignorare il tasso di occupazione del Sud, per cento, contro il 70 per cento del Settentrione. E ancora, vorrebbe dire ignorare che l'indice della disoccupazione giovanile al Sud è il terzo più alto dell'Unione europea. Perciò mi chiedo e vi chiedo: ha senso parlare di costo della vita, quando chi nasce nella mia terra è già soggetto a una tassa occulta, che lo rende un cittadino di serie B? Ragion per cui, solo dal 2002 al 2017, oltre due milioni di cittadini hanno abbandonato il Mezzogiorno, più della metà giovani, il 33 per cento Presidente, solo altre due parole. Onorevoli colleghi della maggioranza, sul tema ho depositato un'interrogazione parlamentare, perché non vi posso consentire di tenere in ostaggio il futuro dei nostri figli, su cui non deve ricadere la vostra bulimia partitica. Pertanto, anche se è questo il vostro obiettivo, il MoVimento 5 Stelle non vi consentirà di gettare le basi per la secessione. Grazie per l'attenzione.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

si celebrava e purtroppo si commemorava il colpo di stato che in Myanmar ha riportato al potere una giunta militare feroce e una dittatura contro cui il popolo birmano si sta battendo. Due anni che appunto non hanno cancellato la tenace e coraggiosa resistenza di un popolo, né quella di Aung San Suu Kyi, *leader* della LND, condannata a trentatré sul quale è sceso un oblio davvero inquietante a livello internazionale. Né sono venute meno la capacità e la voglia di resistenza dei parlamentari e delle parlamentari

avuto l'opportunità e l'onore di svolgere un incontro in videocollegamento con alcune donne parlamentari alla macchia, dalle cui voci abbiamo appreso la drammaticità della situazione del popolo, ma anche il bisogno e la speranza, che nutrono e che coltivano, della vicinanza della comunità internazionale. Soltanto ascoltandole, si comprende quanto per loro sia importante sentire vicina la comunità internazionale. L'oblio che sembra invece sceso sul dramma di quel Paese e di quel popolo per fortuna è stato recentemente che provengono da più parti del mondo a livello internazionale. Cina, Russia e India non si sono opposte alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che chiede il ritorno alla democrazia per la Birmania. Anche l'ASEAN ha insistito per il cambiamento politico del Myanmar. L'Italia e l'Unione europea (che in passato ha giocato un ruolo davvero importante nella richiesta di liberazione dalla prima prigionia di Aung San Suu Kyi nominando un inviato speciale per la Birmania), continuano a sostenere un nuovo avvio del processo di democratizzazione di quel Paese. Noi da qui, dal Senato, vogliamo semplicemente rivolgere a quel popolo le seguenti parole: "Noi siamo con voi, al fianco di ogni donna e di ogni uomo che combatte per la libertà e la democrazia. La vostra battaglia è la nostra battaglia. Il vostro sogno è il nostro sogno". Voglio concludere con le parole di Aung San Suu Kyi, in una sorta di preghiera per il suo popolo: "Ciascuno di noi sia un rifugio sicuro per la democrazia".